Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia:* «Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena»

29 giugno è scomparsa a Trieste, all'età di 91 anni, la professoressa Margherita Hack, astrofisica di fama internazionale. Nata a Firenze il 12 giugno 1922, nel 1964 divenne titolare della cattedra di astronomia nell'Università degli studi di Trieste. Fu la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia e sotto il suo impulso l'attività di ricerca dell'osservatorio triestino conquistò la notorietà e l'apprezzamento unanime della comunità scientifica internazionale. Componente dell'Accademia nazionale dei Lincei e di numerose istituzioni e gruppi di lavoro internazionali, era nota a tutti gli italiani grazie alla sua instancabile attività di divulgazione scientifica. Grazie ai suoi scritti, interviste e partecipazioni televisive, Margherita Hack ha ampliato la diffusione e la conoscenza dei grandi temi dell'astronomia e dell'astrofisica anche ad un pubblico non accademico. La sua tenacia e la sua passione per la ricerca furono una testimonianza coerente delle ragioni e degli ideali del sapere scientifico, da lei interpretata come un vero e proprio impegno civile. Tale impegno si radicava nella fiducia che gli strumenti della scienza permettessero di comprendere le origini e i meccanismi di funzionamento dell'universo. Fiducia significava per lei non tanto facile ottimismo quanto piuttosto costanza, rigore e serietà nella ricerca scientifica. Nel suo ultimo volume vi è il segno del suo tratto esigente e allo stesso tempo consapevole dei limiti dell'approccio scientifico: la scienza spiega il come, ma non il perché della vita. Dalla consapevolezza delle potenzialità e dei limiti della scienza originava la sua prospettiva di scrivere dentro il perimetro sociale il proprio percorso scientifico Margherita Hack viveva come inscindibili i due piani, soprattutto per la promozione e la difesa dei diritti fondamentali. Aveva anche accettato più volte di candidarsi in occasione di elezioni politiche, europee, regionali e locali, ma sempre rinunciando al seggio. Negli ultimi mesi il suo impegno sociale era tornato a concentrarsi sulle ragioni della ricerca italiana, in particolare dei giovani ricercatori, con un appello a favore di una maggiore stabilità e valorizzazione del loro lavoro riconsiderando in particolare la scelta di abolire i contratti a tempo indeterminato per quanti scelgono di dedicare la propria esistenza alla ricerca scientifica. Il suo coraggio e la sua determinazione per sostenere i giovani, per aprire loro ogni possibilità di crescita e di avanzamento fondata sul merito, il più delle volte proprio a loro preclusa, aprirono la sua scuola ben oltre le aule universitarie. La sua scuola divenne una vera e propria comunità dei saperi. Sono certo di interpretare il sentimento commosso di tutto il Senato nel manifestare il cordoglio e la partecipazione della nostra Assemblea al dolore della famiglia di Margherita Hack, e in particolare del marito Aldo De Rosa, suo compagno di vita per quasi settant'anni, nonché dei colleghi e degli allievi nella comunità scientifica italiana ed internazionale. Invito quindi i colleghi ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento in memoria di questa grande figura di donna e scienziata.

Scienziata chiarissima a cui l'Osservatorio astronomico di Trieste, di cui fu direttrice per oltre vent'anni, deve la sua meritata fama internazionale, non considerò mai la scienza come qualcosa di diverso e separato dall'impegno sociale e dal rigore etico, e nel riconoscere e affermare il suo limite rimarcava ancora di più quanto fossero necessari un fondamento ed un rigore etico nell'approccio scientifico. Al contrario, proprio perché era una scienziata, riusciva sempre a considerare la realtà nella sua completezza. Si batteva allo stesso modo in difesa della giustizia sociale e dell'ambiente.

L'abbiamo avuta a fianco in tante battaglie a difesa degli animali perché per lei tutto ciò che viveva doveva essere difeso.

Non c'era quasi differenza fra i suoi grandi amori, l'astrofisica e i suoi gatti, perché in entrambi i casi si trattava di schierarsi a favore della vita, della cultura, contro le forze e le logiche che minacciano entrambi. La scienza mondiale scrive il nome della Hack accanto a quello dei grandi ricercatori che hanno tenuto alto tra gli Stati il prestigio scientifico italiano. Lascia un vuoto enorme nella cultura italiana poiché è stata un punto di riferimento per molti di noi. Lo sarà - io spero - anche per i nostri figli e per le generazioni future.

Margherita Hack è stata una delle menti più brillanti della scienza astrofisica mondiale. Prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia, ha dato un considerevole contributo alla ricerca per lo studio e la classificazione di molte categorie di stelle. Era nata in una famiglia in cui il padre, di religione protestante, e la madre, di religione cattolica, entrambi critici e insoddisfatti della propria appartenenza religiosa, aderirono alle dottrine che propugnano la fratellanza universale dell'umanità, incoraggiano lo studio comparato delle religioni, filosofie e scienze, e investigano sulle leggi inesplicate della natura. Forse per questo la Hack fu attratta dallo studio della natura e delle leggi che la regolano.

Nel 1945, finita la guerra, Margherita Hack si laurea in fisica a Firenze con una tesi di astrofisica. Nel 1954 ottiene la libera docenza e inizia la sua attività di divulgatrice scientifica, collaborando con importanti riviste. È proprio in questa attività che la Hack eccelle, riuscendo a far capire a tutti, in modo semplice, le leggi che regolano l'universo, utilizzando esempi di immediata comprensione. Ha alternato, infatti, la stesura di testi scientifici universitari alla scrittura di testi a carattere divulgativo. Il trattato «Stellar spectroscopy», scritto a Berkeley nel 1959, è considerato ancora oggi un testo fondamentale nel settore. Collabora con prestigiose università straniere e nel 1964 diviene professore ordinario, ottenendo la cattedra di astronomia presso l'Istituto di fisica teorica dell'Università di Trieste. In qualità di professore ordinario assume l'incarico della direzione dell'Osservatorio astronomico. La sua gestione durerà per più di vent'anni, fino al 1987, e darà nuova linfa a un'istituzione che in Italia era ultima sia per numero di dipendenti e ricercatori sia per qualità della strumentazione scientifica, arrivando a darle risonanza anche in campo internazionale.

Nel 1992 ha terminato la carriera di professore universitario, continuando, tuttavia, l'attività di ricerca, dedicandosi a incontri e conferenze al fine di diffondere la conoscenza dell'astronomia e una mentalità scientifica e razionale. Politicamente molto impegnata, è stata iscritta all'Associazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca scientifica e al Partito Radicale Transnazionale, anche se tutte le volte che aveva scelto di impegnarsi in prima persona si era candidata sempre con partiti di sinistra. Era atea convinta, non credeva in nessuna religione o forma di soprannaturalismo. Riteneva inoltre che l'etica non derivasse dalla religione, ma da «principi di coscienza» che permettono a chiunque di avere una visione laica della vita. Pur non condividendo alcune sue esternazioni, spesso pungenti nei confronti dei suoi avversari, rispettiamo la forza d'animo e la convinzione con cui ha sempre cercato di far comprendere il suo pensiero. La Lega Nord si associa nell'espressione di sentimenti di profondo cordoglio ai familiari della scienziata, della quale, oltre ad apprezzare l'indubbia eccellenza nell'attività di divulgazione scientifica, condivide in pieno il suo impegno nella difesa delle lingue dei popoli, contraria come era all'utilizzo esclusivo ed obbligatorio della lingua inglese per l'insegnamento delle materie scientifiche nelle università italiane. «Secondo me» - diceva - «non bisogna abbandonare la propria lingua, certi concetti si possono esprimere solo quando una lingua si conosce molto bene come la propria».

Margherita Hack aveva compiuto da pochi giorni 91 anni quando si è spenta, come avete ricordato, nella sua Trieste d'adozione, dopo avere diretto, prima donna, per oltre trent'anni, l'Osservatorio astronomico. 91 anni sono gli stessi che avrebbe compiuto mia madre se fosse ancora in vita e gli stessi che sono trascorsi dall'inizio delle celebrazioni in Italia della Festa della donna. donna. Quasi un secolo, quindi, drammaticamente attraversato dalla tragedia della guerra, ma anche dalle più rapide e sconvolgenti rivoluzioni tecnologiche e scientifiche che l'umanità avesse mai conosciuto, come la Hack amava ricordare nelle poche, pochissime riflessioni dedicate al passato

Quella generazione di donne - forse è bene ricordarlo anche oggi - aveva attraversato almeno tre grandi rivoluzioni nel Novecento, come figlie, come mogli e come madri: come figlie, al ritmo dei nuovi balli americani del dopoguerra e per pochissime, veramente pochissime, con l'ingresso consentito nelle facoltà universitarie, nelle professioni e nel mondo della ricerca; come mogli, nell'impegno quotidiano come operoso e incessante contribuito alla ricostruzione del Paese e alla sua incredibile ripresa fuori e dentro casa; come madri, infine, di noi figli e figlie degli anni Sessanta, educate a diventare donne in una società più libera e avanzata. Ma la Hack era una donna molto speciale. Una punta di diamante, mi verrebbe da dire, di quella generazione; anomala e stravagante per natura e per cultura; astronoma quasi per caso, ma scienziata per dedizione verso quell'unica religione cui lei riconosceva fondatezza e autorità: la ragione, la scienza e il costante bisogno di conoscenza. Su questa base la signora delle stelle ha combattuto una battaglia quotidiana, intellettuale e politica contro i suoi veri antagonisti: la superstizione e l'ignoranza prima di tutto, ma anche la rassegnazione ad un declino culturale apparentemente senza rimedi che le pareva insopportabile. Il suo testamento spirituale, che si desume dai molti scritti, anche solo dai titoli di questa sterminata bibliografia, è eterogeneo ma comunque percorso da un pensiero coerente. Lo riassumo con le sue parole: «Ho attraversato un secolo con la voglia di vincere». E questa energia Margherita Hack l'ha portata in tutti i campi dell'esistenza: dalla carriera accademica al dibattito politico e culturale, anche alla vita quotidiana, quella privata. Ricordo che quando le fu tolta la patente per raggiunti limiti di età, età, con toscanità incontenibile protestò dicendo che aveva una Panda, dal 1952 guidava dappertutto, non aveva mai avuto gravi incidenti e quindi il comportamento del medico era assolutamente incostituzionale. Hack il tema dominante era l'idea che una società più istruita sarebbe stata anche più coraggiosa, anche più visionaria e quindi una società migliore. E con questa lucidità non ci stava a veder crollare il suo Paese, né risparmiava ai potenti che lo guidano e che lo guidavano lo stimolo e la provocazione. Ai ragazzi, allievi diretti e ormai non più diretti, ha rivolto di recente un suggerimento chiaro e semplice che vorrei fossimo in grado di dare ai nostri studenti nelle università: scegliete la professione che vi interessa di più; quando dovete decidere cosa studiare non pensate solo a quello che vi permetterà di trovare un lavoro, ma a quello che vi piace veramente. E alle ragazze, in particolare, dico di avere più fiducia in se stesse, pretendere che i loro diritti vengano rispettati e, da ex sportiva, aggiungo affrontate la vita come una gara, con la voglia di vincere.

E del futuro del nostro Paese si preoccupava nel dettaglio, perché è inutile parlare di innovazione e di ricerca se si taglia sempre e soprattutto lì, perché è persino ipocrita continuare a predicare la religione della scienza e della cultura senza che da ciò derivi un preciso e incrollabile impegno a mettere al centro delle agende politiche dei Paesi avanzati questo tema. tema. A noi oggi, cari colleghi, figli e figlie di madri silenziosamente rivoluzionarie, sicuramente più silenziose di Margherita Hack, ma della stessa generazione, resta soprattutto questo compito urgente e complesso nella cultura e nella società italiana, ricordando questa straordinaria, eccezionale figura.

*(M5S)*. Signor Presidente, il Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle si associa al cordoglio unanime espresso per la scomparsa della professoressa Margherita Hack, il volto più noto dell'astrofisica italiana. Vogliamo ricordare innanzi tutto la sua brillante carriera professionale. È stata autrice di oltre 200 pubblicazioni, come prima autrice, e sulle più prestigiose riviste specializzate. Sottolineiamo, tra i tantissimi contributi, quelli sulle variabili cefeidi, uno dei primi gradini della scala di misurazione delle distanze cosmiche, e quelli sulle stelle binarie variabili cataclismiche, affascinanti sistemi di stelle doppie in cui una stella risucchia il materiale dell'altra causando enormi esplosioni termonucleari. Il Presidente ha già ricordato il suo impegno presso l'Osservatorio di Trieste, per il rilancio di questa struttura che oggi appartiene all'Istituto nazionale di astrofisica. Vogliamo inoltre sottolineare le sue qualità umane e di grande comunicatrice dei nostri tempi. Margherita Hack è stata impegnata in tutta la sua vita in attività di divulgazione scientifica per avvicinare il mondo della ricerca astronomica al grande pubblico. Ricordiamo la fondazione della rivista "L'Astronomia" e i tanti libri che ha scritto proprio per avvicinare il pubblico alla materia. Con la scomparsa di Margherita Hack esce di scena una delle più autorevoli voci a sostegno della ricerca scientifica, una voce che ha sempre difeso la ricerca, l'università e l'istruzione dal modo in cui sono state trattate negli ultimi anni. Era - non dimentichiamolo - una voce laica, che ha sempre difeso la scuola pubblica e la necessità di rispettare il dettato costituzionale circa il finanziamento alle scuole private. Era una voce per il rispetto del diritto degli animali, com'è stato ricordato. Era anche una voce con un inconfondibile accento fiorentino, che sono sicuro ora tutti ricordiamo e quasi sentiamo nelle nostre orecchie, con il quale comunicava simpatia, ma anche fermezza e determinazione. Instancabile ed indomabile, Margherita Hack, fino agli ultimi giorni della sua vita, anche quando le sue condizioni di salute non erano più ottimali. 5 Stelle, di cui mi onoro personalmente di far parte, ed il grande pubblico la ricordano sempre disponibile ad intervenire, anche se ormai non di presenza, a convegni, dibattiti ed interviste. Il Movimento 5 Stelle, pur nella diversità di alcune vedute, ma nel rispetto pieno delle sue opinioni, vuole raccogliere il suo messaggio facendosi anch'esso portatore di un'idea nuova di società, in cui l'istruzione e la ricerca siano volano di crescita individuale e collettiva. I fondi ad esse destinati non devono essere classificati come semplice spesa, cari colleghi, ma come veri investimenti nel capitale umano. Grazie, Margherita, adesso sei anche tu una stella in quel firmamento che tanto hai amato e divulgato.

è scomparsa Margherita Hack e scompare l'icona del pensiero libero e dell'anticonformismo, come l'ha definita assai bene Umberto Veronesi. Ma la signora delle stelle era anche altro: oltre l'impegno scientifico che l'ha resa famosa in tutto il mondo, oltre l'impegno politico nella sinistra più laica e radicale, la ricordiamo anche per un'altra vita iniziata a novant'anni, quella che lei racconta tra confessioni, sorrisi, bilanci e progetti, riflessioni condivise con don Pierluigi Di Piazza, prete di strada, in quel mirabile confronto tra il diavolo e l'acqua santa cominciato vent'anni prima e raccontato nel libro «Io credo»: un esempio di come l'etica, l'impegno, la scienza e la conoscenza aperta al prossimo e alla società siano un reale punto di partenza verso nuovi orizzonti, che fanno del rispetto e dell'ascolto il loro credo, nel segno del progresso civile, nel rispetto per tutti gli esseri viventi, dell'accoglienza, della coerenza e dell'impegno costante. Nata in quella Mitteleuropa delle piccole patrie ma cittadina del mondo, la ricordiamo per le efficacissime interviste dalla sua casa, quella animata dal suo sorriso, dove si respirava aria di libertà, di scienza e di conoscenza, circondata dai libri (una biblioteca di 24.000 volumi), suo marito, gli otto gatti e un cane. La vogliamo ricordare così anche oggi, oggi che Marghe è salita tra le sue stelle, quelle che tante volte ci ha raccontato e ci ha insegnato a capire e forse ad amare come lei. Signor Presidente, lo hanno riportato molti colleghi i quotidiani di tutto il mondo l'hanno ricordata come la signora delle stelle. Era l'icona e il riferimento dell'astrofisica mondiale. Come ha dichiarato il presidente Napolitano, è stata personalità di grande rilievo del mondo della cultura scientifica. Con i suoi studi e il suo impegno di docente ha costantemente servito e onorato l'Italia anche in campo internazionale, ma allo stesso tempo ha rappresentato un forte esempio di passione civile, lasciando un'impronta nel dibattito pubblico e nel dialogo con tutti i cittadini.

e, parlandoci dei suoi primi novant'anni (così li ha raccontati nel libro «Nove vite come i gatti»), ci ha detto di quanto fossero stati fondamentali nella sua vita e nella sua formazione i suoi genitori, babbo protestante e mamma cattolica, entrambi poco poco soddisfatti della propria religione (così ce li raccontava con le sue parole), che l'avevano educata alla teosofia. Da ragazza era stata anche un'atleta di valore e ricordava con orgoglio di aver vinto due campionati universitari di salto in alto e di salto in lungo, ma soprattutto non aveva mai abbandonato la sua passione per la bicicletta. All'emanazione delle leggi razziali era diventata immediatamente antifascista e considerava il razzismo come uno degli orrori più gravi dell'umanità. atea, considerava tutti fratelli della stessa zuppa primordiale che proviene dal Big Bang, e per questo il suo credo era innanzitutto un profondo rispetto per tutti gli esseri umani e per gli animali. Era infatti anche, come avete ricordato, vegetariana e convinta animalista, ma soprattutto nella vita la guidava - ci aveva raccontato quella sera - il credo etico che recita «non fare mai agli altri quello che non vorresti fosse fatto fatto a te». Da donna e studiosa appassionata invitava i giovani a seguire le proprie inclinazioni, a fare ciò che piace, ma con serietà ed impegno. Considerava però sciocco - ci aveva detto - invitare i giovani a cambiare spesso lavoro poiché, invece, era convinta che nel lavoro servano specializzazione e approfondimento. Era profondamente rammaricata per le tante intelligenze e i tanti giovani talenti costretti ad abbandonare il nostro Paese, lo considerava masochistico sperpero di risorse. Li formiamo bene - ci aveva detto - nelle nostre ottime università ma poi, non investendo nella ricerca, lasciamo che i migliori ricercatori vengano valorizzati da altri Paesi, che così beneficiano dei nostri investimenti. Ci ricordava

un calcolatore elettronico, l'ELEA, e il primo *personal computer*, con l'Olivetti. E poi, appunto, quella grande azienda, quel grande patrimonio è stato perso con poca lungimiranza per aver smesso di investire in ricerca ed innovazione. È stata soprattutto, come lei ha ricordato, Presidente, una straordinaria divulgatrice scientifica. Ci diceva che riteneva la divulgazione scientifica un dovere morale per uno scienziato, che serve ancora di più a chi la fa che a chi la riceve, perché, per spiegare con parole semplici la scienza, occorre prima capire molto bene i concetti

testamento spirituale. Al marito Aldo, a cui è stata legata per settant'anni, a tutta la comunità scientifica e ai suoi allievi vanno le più sincere ed affettuose condoglianze del Partito Democratico. Nella seduta antimeridiana di oggi l'Assemblea ha ricordato il 4° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto presso la stazione di Viareggio il 29 giugno 2009, nel nel quale persero la vita 33 persone. La Presidenza si associa alle parole di cordoglio e di commemorazione delle vittime del tragico evento e invita l'Assemblea ad un minuto di raccoglimento.

Invito il senatore Segretario a dare lettura della comunicazione pervenuta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

le ha dichiarate valide: Vito Rosario Petrocelli e Guido Walter Cesare Viceconte; per la Regione Calabria: Pietro Aiello, Giovanni Emanuele Bilardi, Antonio Stefano Caridi, Vincenzo Mario Domenico D'Ascola, Antonio Gentile, Doris Lo Moro, Domenico Minniti, Francesco Molinari, Nicola Morra e Domenico Scilipoti; per la Regione Liguria: Donatella Albano, Massimo Caleo, Cristina De Pietro, Paolo Guerrieri Paleotti, Augusto Minzolini, Roberta Pinotti, Maurizio Giuseppe Rossi e Vito Vattuone; per la Regione Marche: Silvana Amati, Remigio Ceroni, Camilla Fabbri, Serenella Fucksia, Maria Paola Merloni, Mario Morgoni, Riccardo Nencini e Francesco Verducci; per la Regione Piemonte: Alberto Airola, Daniele Gaetano Borioli, Enrico Buemi, Vannino Chiti, Michelino Davico, Nerina Dirindin, Stefano Esposito, Nicoletta Favero, Elena Ferrara, Elena Fissore, Federico Fornaro, Stefano Lepri, Lucio Malan, Patrizia Manassero, Mauro Maria Marino, Carlo Martelli, Andrea Olivero, Manuela Repetti, Maria Rizzotti, Marco Scibona, Gianluca Susta e Magda Angela Zanoni; per la Regione Sardegna: Alessandra Bencini, Laura Bottici, Laura Cantini, Rosa Maria Di Giorgi, Valeria Fedeli, Marco Filippi, Maria Grazia Gatti, Stefania Giannini, Manuela Granaiola, Andrea Marcucci, Claudio Martini, Altero Matteoli, Donatella Mattesini, Riccardo Mazzoni, Sara Paglini, Alessia Petraglia, Maurizio Romani e Denis Verdini; per la Regione Trentino-Alto Adige: per la Regione Umbria: Valeria Cardinali, Nadia Ginetti, Miguel Gotor, Linda Lanzillotta, Stefano Lucidi, Gianluca Rossi e Luciano Rossi; per la Regione Valle d'Aosta: Albert Lanièce.

recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il mio intervento è legato alla necessità di sostenere, in ogni modo possibile, le aziende, e (in particolare l'industria dell'elettrodomestico, che stanno rispondendo al rapido decrescere del fatturato con licenziamenti e delocalizzazioni. Nella relazione illustrativa al provvedimento l'altro, che la disposizione intende favorire la ripresa economica e l'offerta occupazionale nel settore legno, attualmente in forte crisi; tuttavia anche il settore industriale degli elettrodomestici *made in Italy*, secondo comparto manifatturiero in Italia dopo quello dell'automobile, che occupa oltre 130.000 lavoratori, è da tempo alle prese con una difficile situazione. In particolare, dal 2002 al 2012 si è registrato un dimezzamento dei volumi di produzione, passati da 30 milioni di pezzi Nell'ultimo triennio, dal 2010 al 2012, le imprese del commercio hanno visto decrescere il proprio fatturato legato alla vendita

nel primo trimestre del 2013, il fatturato è sceso di oltre il 15 per cento. A questo si aggiunga la stima dei possibili licenziamenti annunciati anche da grandi aziende, tipo l'Electrolux, che prevede ben 1.129 esuberi in vari stabilimenti italiani, nonché la ormai nota vicenda Indesit, i cui vertici aziendali hanno annunciato un piano di ristrutturazione che interesserà tre siti italiani (quello di Fabriano, in provincia di Ancona, quello di Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno, e quello di Caserta), ridisegnando completamente la loro missione strategica con la concentrazione nel nostro Paese delle sole produzioni di *top* di gamma e lo spostamento delle produzioni italiane nei siti Indesit in Polonia e Turchia. A tale riassetto produttivo si accompagnerà una razionalizzazione delle risorse umane che, secondo quanto annunciato dai vertici aziendali, coinvolgerà complessivamente 1.425 lavoratori. Quanto detto, aggiunto alla ridotta capacità di spesa da parte dei cittadini e al rischio di non poter nemmeno più detrarre le spese sostenute per l'acquisto di elettrodomestici, configura uno scenario più che preoccupante per l'economia attuale e futura. È proprio a questo proposito che ho presentato l'ordine del giorno G16.103, in cui la combinazione delle varie proposte fatte al Governo allo scopo di sostenere il mercato dell'elettrodomestico italiano dovrebbe avere una notevole ricaduta positiva su tutta la filiera. In riferimento al predetto ordine del giorno, vorrei, anzi, chiedere se sia possibile integrarlo con due altri punti d'impegno da parte del Governo: la previsione di incentivi ai soli elettrodomestici almeno A+ A+ prodotti in Italia, e l'estensione di quanto previsto per gli acquisti anche alle abitazioni secondarie, studi, uffici e quant'altro. Chiedo, quindi, se sia possibile una riformulazione in tal senso dell'ordine del giorno. Ribadisco l'importanza che rivestono tutte queste azioni per non vedere sparire tante aziende italiane, anche grandi e di lunga tradizione, fortemente colpite dalla crisi con delle ripercussioni e dei danni anche a più lungo termine forse ancora maggiori. Ricordo che dietro un'azienda ci sono i drammi di molte famiglie, di famiglie intere e di persone che, perdendo il lavoro, subiscono non solo un danno economico, ma di motivazione, autostima e - brutto a dirsi - di dignità. Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, non possiamo che salutare con favore l'approvazione del decreto-legge al nostro esame, che recepisce, attraverso le modifiche e le integrazioni alle disposizioni contenute nel decreto-legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la direttiva europea 31 del 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, prorogando e potenziando al contempo incentivi fiscali di grande importanza previsti per il miglioramento dell'efficienza energetica in edilizia. Questo provvedimento servirà a mettere la parola fine alla procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea il 24 settembre scorso, proprio per il mancato recepimento di quella direttiva, e a porre definitivamente rimedio anche ad un'altra procedura d'infrazione aperta dalla stessa Commissione il 18 ottobre 2006, a causa del parziale e non conforme recepimento della direttiva n. 91 del 2002. La finalità della direttiva comunitaria del 2010 è coerente con l'obiettivo di raggiungere la riduzione del 20 per cento delle emissioni di CO2 entro il 2020, in un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione europea. tenuto conto delle condizioni locali e climatiche esterne, promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione, e detta prescrizioni riguardo al clima degli ambienti interni e all'efficacia anche sotto il profilo dei costi. La prima parte del provvedimento è diretta a modificare il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per adeguarlo a quanto previsto dalla direttiva del 2010: le disposizioni in esso contenute si muovono nella giusta direzione che è quella, cioè, di dare maggiore

sostituendo alla certificazione energetica quella di prestazione energetica, cui si ricollega una metodologia di calcolo che dovrà risultare da una serie di atti attuativi, previsti in particolare dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge al nostro esame. A questo proposito vorrei rivolgere un invito a tutte le colleghe e i colleghi ad accogliere l'emendamento da noi proposto, che prevede una specifica clausola di salvaguardia che permette alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alle Regioni a Statuto speciale di risolvere i problemi applicativi nella fase di transizione da parte loro c'è già stato un parziale recepimento della direttiva precedente. Qualche perplessità rimane sull'entità delle sanzioni, piuttosto elevate, previste a carico del proprietario o del conduttore dell'unità immobiliare che non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione; nonché quelle a carico del responsabile dell'annuncio commerciale di offerta in vendita o locazione dell'immobile che viola l'obbligo di riportare nello stesso i parametri energetici: sanzioni che a nostro avviso andrebbero ridimensionate. La seconda parte del provvedimento contiene diverse misure, molto attese, che produrranno un impatto positivo sugli investimenti e sui consumi nel settore immobiliare; come il cosiddetto ecobonus, ossia l'agevolazione fiscale del 65 per cento, prevista per le spese documentate

dicembre 2013 della maggiore detrazione IRPEF, dal 36 per cento al 50 per cento, e del limite dell'ammontare complessivo detraibile, da 48.000 a 96.000 euro, in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia. Tali agevolazioni, che ci auguriamo possano celermente entrare a regime, hanno riscosso negli anni passati notevole successo e aiutato molte famiglie ed aziende ad affrontare spese altrimenti non sostenibili in un periodo di grande crisi come quello che stiamo attraversando. L'*iter* del provvedimento, assegnato alle Commissioni riunite 6a e 10a, è stato comunque complesso. Sono state molte le proposte di modifica presentate al testo, alcune condivisibili, perché dirette a sciogliere alcuni nodi evidenziati nel provvedimento, ma che per evidenti ragioni di copertura finanziaria non hanno potuto trovare accoglimento. Mi riferisco in particolare a quegli emendamenti che proponevano di includere nell'ecobonus alcuni impianti considerati tra quelli volti a garantire un elevato risparmio energetico, come le pompe di calore ad alta efficienza o gli impianti geotermici a bassa entalpia. Ci auguriamo a questo proposito che il Governo tenga comunque presente quanto emerso in sede di dibattito nelle Commissioni di merito per riportare appena possibile nel regime delle agevolazioni anche questi impianti. Vogliamo esprimere il nostro apprezzamento per la positiva convergenza di tutti i membri delle Commissioni riunite sulle proposte di modifica intese ad allargare anche agli elettrodomestici di classe A+

Desidero anche, personalmente, ringraziare il Governo per aver recepito con l'articolo 17 del provvedimento al nostro esame quanto richiesto con 1'interrogazione parlamentare 3-00045 riguardante la qualificazione degli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili. La disposizione consente agli operatori del settore che hanno lavorato per almeno tre anni in qualifica di operaio specializzato di continuare, anche dopo il 1° agosto 2013, la loro attività di installatori di pannelli solari o fotovoltaici, a biomasse, solari termici, pompe di calore e geotermici, permettendo così a circa 80.000 imprese italiane attualmente in attività di poter continuare ad operare in uno dei pochi settori di mercato che mostra ancora potenzialità di crescita. In conclusione, la nostra valutazione in generale sul provvedimento è positiva, anche se alcune disposizioni relative alla copertura degli oneri previsti dal decreto-legge ci lasciano perplessi, in quanto potrebbero avere un ricaduta negativa sul settore dell'editoria e più in generale sulla cultura. Il rilievo riguarda, in questo caso, la modifica della disciplina dell'IVA riguardante le cessioni di prodotti editoriali, che dal 1° gennaio 2014 prevede un aumento dell'aliquota dal 4 per cento al 21 per cento. Ad essere colpiti da questo aumento non sono solo i *gadget* allegati alle pubblicazioni, ma anche i «beni funzionalmente connessi» ai libri e ai periodici, ovvero quelli che ne rappresentano il completamento

È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

Avremmo potuto e voluto fare di più, all'interno delle Commissioni, e avremmo voluto e potuto contribuire a un miglioramento ulteriore, così come altri colleghi hanno già sottolineato.

Ci sono dei punti di forza che vanno evidenziati. In primo luogo si adempie finalmente a una direttiva europea di alto valore etico, che persegue lungimiranti obiettivi sociali ed economici:

Questi provvedimenti, infatti, aiuteranno sicuramente le imprese, i produttori e gli artigiani. Il terzo punto di forza

Ebbene, con questo decreto diciamo alle famiglie italiane: dopo aver acquistato la casa, non abbandonatela, miglioratela, aumentate il potenziale di qualità della vostra abitazione. con il provvedimento si combatte anche l'evasione fiscale, perché sì, caro cittadino, cara famiglia, ti diamo il *bonus* fiscale, ma tu metti in chiaro, metti in trasparenza i lavori che farai. Questi sono punti di forza indubitabili,

presentato in tal senso come una breve pausa di riflessione, in attesa che venga invece ripresa un'attenzione seria sul problema degli adeguamenti sismici, che non sono meno importanti dell'efficientamento energetico.

che deve affrontare questo tema; non può rinviarlo ogni volta e sempre. In questi giorni nella Lunigiana ci sono popolazioni afflitte dalla paura. Se fossimo sicuri che le scuole, le case, gli uffici corrispondano a requisiti di sicurezza non ci sarebbe la necessità di evacuare, di organizzare tendopoli, di mettere in fibrillazione intere popolazioni e la loro economia. Ecco quindi che rilancio, con il Gruppo del Partito Democratico e con altri Gruppi che pure intendevano sostenere l'esigenza di affrontare questa questione, la necessità di prevedere altri incentivi e sistemi di aiuto a quelle famiglie e a quegli enti locali che intendono mettere in sicurezza il proprio patrimonio dal punto di vista del rischio sismico. È inutile altrimenti piangere ogni volta lacrime di coccodrillo;

Per l'Emilia-Romagna serviranno molte risorse, ne serviranno tantissime per l'Abruzzo, ne sono servite tante per il Belice, per l'Irpinia e per il Friuli. Quanto, invece, costerebbe mettere in sicurezza il nostro Paese? Sicuramente tanto, ma se non si inizia mai non avremo mai case, scuole,

di riflessione di quest'Aula e del Governo, che ha accompagnato questo provvedimento. Parlo di un patrimonio di riflessione e di bisogno profondo di dare una risposta per non essere il Paese delle lacrime di coccodrillo, ma il Paese che mette in sicurezza il proprio patrimonio e che consente agli enti locali, anche attraverso interventi sul Patto di stabilità, di poter mettere anch'essi in efficienza, oltre che energetica, anche antisismica, il proprio patrimonio Credo che il decreto abbia una sua forza: ci permette di investire sull'economia collegata all'efficientamento energetico e e alla cosiddetta economia verde; ci consente insomma di ammodernare il nostro Paese dando lavoro, e credo che questo sia un obiettivo prioritario del Governo e della maggioranza: sicuramente lo è del Partito Democratico. Possiamo aprire altre riflessioni. Tutte le categorie che hanno partecipato alle audizioni hanno sottolineato quanto il nostro patrimonio urbanistico ed edilizio sia vetusto. La gran parte delle abitazioni risale a prima del 1971, ovvero a prima delle norme e della legislazione che prevede degli *standard* di sicurezza più adeguati. Questo significa che abbiamo un territorio, delle abitazioni e degli edifici ancora insicuri. Interveniamo anche con la leva fiscale, visto e considerato che altri sistemi hanno difficoltà ad essere approntati a causa della grave crisi dell'economia, ma facciamolo. Lo prendo Lo prendo come un rinvio, però chiedo un impegno del Governo su questa necessità del Paese.

però mi consenta di dire - mi rivolgo soprattutto al rappresentante del Governo - che voglio considerare questo provvedimento solo come un primo passo. L'Italia, infatti, è in grave ritardo, un ritardo non solo nei confronti della Commissione europea, ma un ritardo, prima di tutto, di carattere culturale. introdurre l'efficienza energetica e fare un ragionamento sulle fonti naturali e su tutte le altre novità contenute in questo decreto-legge vuol dire ripensare un settore, quale appunto quello edilizio, di primaria importanza, perché ha permesso di produrre ricchezza e benessere, facendo da traino a tanti altri settori e generando uno sviluppo senza precedenti. E allora questo provvedimento oggi ci permette di sanare almeno in parte questo ritardo culturale: pensare che lo sviluppo può essere considerato tale solo quando è sostenibile per l'ambiente, solo quando non genera sprechi, solo quando tiene conto dell'impatto che ha sul territorio e solo quando mette le persone nella condizione di poter vivere bene. bene. Ne consegue che affrontare il tema dell'efficienza energetica vuol dire affrontare quello del modello di sviluppo e di crescita che si ha in mente per questo Paese. Con il disegno di legge al nostro esame - ripeto - oggi compiamo un primo importante passo, ma mi auguro che il Governo presenti al più presto un vero e proprio piano per il risparmio energetico, da una parte, e per la riconversione o comunque l'efficientamento edilizio del nostro patrimonio, dall'altra. Sono anche convinto che una questione del genere doveva intrecciarsi in maniera molto più forte e coraggiosa con la capacità di produrre ripresa economica. Sono infatti certo che questo decreto-legge consentirà il rilancio di un settore chiave per la nostra economia ma se la missione di questo Governo e la priorità del Paese è oggi la ripresa economica, l'auspicio è che in futuro disegni di legge così strategici si articolino in modo da massimizzare l'efficacia, da far scaturire veri e propri virtuosismi in grado di liberare su ogni livello la nostra economia e permettere così la ripresa. In Commissione ho presentato alcuni emendamenti, che ho riproposto anche in Aula, con l'idea che vadano nella direzione descritta, quella cioè di massimizzare l'efficacia del provvedimento sul fronte del rilancio economico. Non sono stati accolti dal Governo perché comportano

Credo nell'aumento della detrazione d'imposta su alcune tipologie di immobili sia per favorire il rilancio edilizio che per far emergere il sommerso, così come nella riduzione dell'aliquota IVA sulle prestazioni alle categorie svantaggiate, così come in alcune norme che oggi dovrebbero evitare contenziosi con l'Agenzia delle entrate: si eviterebbe così il malcontento che spesso esplode in maniera anche violenta. tutte misure che avrebbero permesso di stimolare in maniera ancora più decisa il mercato, ma a questo punto non può che rimanere l'auspicio che comunque vi sia, in altre forme e in altre sedi, la possibilità di far rientrare Un'ultima considerazione voglio farla su un articolo di questo decreto-legge, precisamente l'articolo 17, del quale peraltro ha già parlato ampiamente il collega Fravezzi, che va a sanare una situazione davvero paradossale. di parlare di come purtroppo in Italia molto spesso si estromettano fette di protagonisti dal lavoro che normalmente svolgono. Ebbene, credo che oggi occorra davvero, accanto ad un maggior coraggio sul terreno degli sgravi per quei settori in grado di produrre nuova ricchezza, ricchezza, lavorare in termini di rimozione di tutti gli ostacoli che rendono difficile la vita ai tanti che quotidianamente si impegnano, che hanno energia e voglia di fare e che possono essere i veri protagonisti per portare l'Italia fuori dalle secche della crisi. Troppe volte il nostro il nostro Paese fa di tutto per mettere lacci e lacciuoli e per bloccare la libera iniziativa. In questo caso si tratta davvero di piccole questioni, perché il nostro sistema è seminato non da grandi ostacoli, ma da tanti minuscoli impedimenti che, per questo, sono più difficili da rimuovere e, soprattutto, sono ancora più invasivi, più rischiosi. Allora, salutando favorevolmente il provvedimento nel suo insieme, l'augurio è che in futuro si possa avere ancora più coraggio e capacità sia per rimuovere gli ostacoli sia per dare sostegni finanziari, magari sotto forma di alleggerimenti del carico fiscale, per quegli ambiti che possono davvero permettere il rilancio del Paese.

atto si può finalmente sperare di far superare all'Italia la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese proprio per il mancato recepimento delle direttive in materia.

di detrazione, ma strumenti che ci consentiranno di raggiungere il massimo degli obiettivi per quanto riguarda la riqualificazione energetica e l'efficientamento. Quindi, non siamo pienamente soddisfatti del fatto che la proroga sull'efficientamento sia stata prevista soltanto (la proroga di un anno, cioè fino al dicembre 2014, è stata accordata solo per i lavori più complessi dei

indicano una strada, che è quella corretta, quella che ci dice con chiarezza di investire in questi settori, nella riqualificazione energetica degli edifici, nella riqualificazione e nella ristrutturazione degli edifici. La collega Pezzopane sottoponeva all'attenzione dei colleghi la questione dell'adeguamento e delle ristrutturazioni per rispondere alla normativa antisismica che rappresenta una vera, grande priorità in questo Paese. Nel porre tali obiettivi,

Signor Presidente, signora Sottosegretario, onorevoli colleghi, all'interno delle diverse disposizioni contenute nel provvedimento oggi in discussione in quest'Aula, la parte più sostanziosa è senza dubbio quella relativa agli interventi finalizzati a migliorare e sostenere la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano. Certo, non vi è dubbio alcuno che una parte consistente di questo patrimonio immobiliare in Italia sia gestito dagli enti pubblici, che non solo ne detengono una parte, ovvero il patrimonio pubblico, ma che, anzi, in diverse modalità gestiscono tale patrimonio. Gli oltre 8.000 Comuni italiani, in tal senso, giocano un ruolo preponderante: non sta forse in capo a loro la pianificazione urbanistica delle città? E non sono forse sempre i Comuni a rappresentare più di altri gli enti pubblici, dove maggiori sono sempre stati gli investimenti di risorse per realizzare opere e beni pubblici? È tuttavia noto a tutti come negli ultimi anni gli enti locali, ed i Comuni in particolar modo, stiano vivendo una grave crisi economica e finanziaria. Manovre economiche draconiane hanno ridotto le loro disponibilità economiche, mentre provvedimenti di chiaro stampo centralista ne hanno profondamente limitato l'autonomia finanziaria, rendendo di fatto impossibile anche l'erogazione ordinaria dei servizi minimi per i cittadini. Non bastasse ciò, da tempo gli stessi Comuni sono soggetti ad un vincolo che impedisce loro, anche a quelli più virtuosi ed efficienti (non sottovalutiamo questo passaggio importantissimo),

rappresenta, infatti, per i sindaci uno stretto pertugio, dove solo in pochi, e sempre in meno, riescono a passare, lasciando sul campo lunghi rallentamenti nei pagamenti alle aziende: le stesse aziende creditrici che, incapaci di attendere tanto, troppe volte sono costrette a chiudere; con le conseguenze sul PIL e sul livello di disoccupazione che voi tutti conoscete. Per questo motivo, il Gruppo della Lega Nord ritiene che mai come oggi, e che proprio all'interno di un provvedimento come questo, finalizzato a sostenere direttamente il rilancio dell'efficienza energetica del Paese e, indirettamente, un settore come quello immobiliare ed edile, profondamente colpito dalla crisi economica, sia necessario, ed anzi auspicabile, che l'Esecutivo preveda di escludere dai vincoli del Patto di stabilità le risorse in conto capitale utilizzate dai Comuni per realizzare opere e sistemi tecnologici finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica negli edifici di proprietà pubblica. Una disposizione in questa direzione avrebbe il doppio vantaggio di migliorare l'attuale patrimonio pubblico immobiliare e, al contempo, di permettere maggiori investimenti degli enti locali in un'ottica di crescita economica ed urbanistica sostenibile. Un segnale certamente importante (che anzi riteniamo doveroso) per un Paese che da tanto, troppo tempo cerca di uscire dalle sabbie mobili di una crisi sempre più pressante. In tal senso, concludo facendo un piccolo riferimento al comparto industriale, fatto da tante piccole e medie imprese, che, se adeguatamente sostenute, possono rappresentare una reale opportunità di crescita per il Paese. Il decreto in esame ha fornito una parziale apertura, prevedendo specifiche detrazioni a favore del comparto edile e dell'industria del mobile, quest'ultimo composto da tante piccole realtà produttive; tuttavia, sarebbe stato più opportuno indirizzare tali interventi a sostegno delle aziende del *made in Italy* e dei prodotti italiani di qualità, oggi fortemente minacciati dall'aggressiva concorrenza dei mercati asiatici. Anche su questo tema avevamo presentato un emendamento che è stato trasformato in ordine del giorno che poi presenteremo.

il provvedimento in esame punta a riqualificare l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano con la proroga ed il potenziamento dei vigenti meccanismi agevolativi; in particolare, reca disposizioni necessarie ed urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE, per evitare l'aggravamento della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Un passo importante, quello adottato da questo Governo per garantire misure di effettiva crescita, nella consapevolezza che, anche attraverso la promozione e lo sviluppo di una politica stabile, sostenibile e di lungo periodo in materia di efficienza energetica, si possa contribuire a dare ossigeno ad un sistema produttivo nazionale che è in deciso affanno e sconta gli effetti negativi di una situazione di forte crisi economica e sociale, anche dal punto di vista occupazionale. Emerge, infatti, in maniera chiara ed evidente come misure di questo tipo, efficaci e di incentivazione, possano dare uno stimolo alla promozione e alla competitività dell'industria italiana e dell'efficienza energetica per il settore residenziale. audizioni svolte è emerso come tale decreto-legge, intervenendo a sostegno di un settore particolarmente rilevante e trainante per l'economia di questo Paese, quello dell'edilizia e delle costruzioni, possa essere positivo per l'intera economia del nostro Paese. Secondo recenti dati forniti da Confindustria il settore, a marzo 2013, una diminuzione del 20,9 per cento rispetto al marzo 2012 in una situazione di crisi crescente; 690.000 sono i dati della disoccupazione in quel settore, in quel settore, che sta soffrendo anche nella compravendita immobiliare e nella locazione. In questa particolare fase congiunturale il settore sconta anche ritardi strategici nella

costruttiva e il miglioramento dell'intera filiera possono sicuramente svolgere un ruolo strategico nell'efficienza energetica e all'interno degli obiettivi europei di sostenibilità. quindi rappresentare per la nostra industria un'opportunità di crescita, anche esterna, un'occasione per rafforzare il proprio posizionamento competitivo sui mercati internazionali. Inoltre, proprio da questo settore deriva un elevato potenziale di risparmio energetico poco sfruttato. A titolo di esempio, in Italia un edificio costruito secondo *standard* di efficienza energetica consente una riduzione dei consumi fino al 70 per cento rispetto ad uno tradizionale. Quindi sarebbe sicuramente un grande beneficio per la nostra bolletta energetica. Ristrutturare e migliorare qualitativamente il patrimonio esistente, sia pubblico che privato, vuol dire anche non continuare vuol dire anche non continuare a consumare territorio che, come sappiamo, negli ultimi anni è stato cementificato più del dovuto. A fronte di un'istanza generale di un loro rafforzamento, le misure incentivanti adottate sono sicuramente di grande auspicio per andare avanti, per ristrutturare il nostro bellissimo patrimonio. Giudico sicuramente molto bene

Non sono costi sostenuti per il caffè ma per il miglioramento e l'efficientamento dei nostri immobili che potranno dare grandi benefici estetici ed economici all'intera collettività. Le famiglie però dovrebbero poter programmare queste spese con serenità e quindi sarebbe utile che questi provvedimenti non fossero provvedimenti *spot* ma strutturali. Anche per le imprese sapere che la detrazione è strutturale le prospetta nell'idea di una ristrutturazione continua e stabile degli immobili strumentali per avere, anche per la parte immobiliare, quell'efficienza che di solito si riserva agli impianti produttivi. Detrarre dai redditi delle somme immesse nel circuito economico non vuol dire solo spesa per uno Stato ma vuol dire tassazione (IVA e IRPEF delle imprese che beneficiano di quel circuito) e, più che altro, vuol dire occupazione uguale a meno cassa integrazione e meno lavoro nero. Sì, perché questo è il grande problema italiano, almeno per le famiglie: se una spesa non posso dedurla, perché pagare l'IVA, che è un costo e invece può diventare un risparmio immediato? la non cultura che porta alla scorrettezza fiscale non può essere giustificata da questa o quella situazione, ma creare quei meccanismi per cui la fatturazione da da fastidiosa tassa diventa uno strumento per migliorare la nostra vita di cittadini e di contribuenti, premiati dallo Stato che contribuiamo a sostenere, sarebbe veramente un grande risultato per noi tutti ed un cambio culturale per il nostro Paese. Ricordiamo che in alcuni Paesi anche la spesa per la *baby sitter* è detraibile. La Commissione bilancio e il Governo si sono prodigati al meglio ma non sono riusciti a trovare la copertura necessaria. Non è colpa di chi deve tenere sotto controllo i conti, perché i numeri sono numeri e noi tutti sappiamo quanto abbiamo dovuto soffrire come Paese per i conti che non erano in ordine, per un debito pubblico lievitato in maniera esponenziale. Ma oggi, alla luce di questa crisi (sarebbe utile ricordare soltanto il tasso di disoccupazione: dato di oggi è il 12,2 per cento) che sta mietendo imprese e posti di lavoro, dobbiamo porci degli obiettivi nuovi, guardare al futuro con prospettive diverse, come farebbe un padre di famiglia o un imprenditore per la propria azienda. Non c'è più tempo, dovremmo avere la forza, e quella purtroppo è una cosa che spetta a noi, a questo Parlamento e al Governo che questo Parlamento sostiene, di fare quelle riforme per eliminare la spesa improduttiva di questo Stato ed investire in quella che produce posti di lavoro, ricchezza, ma soprattutto benessere e libertà. Per fare questo tutti noi abbiamo l'obbligo di mettere da parte le nostre esigenze, personali e di partito, di prestare attenzione a quelle dei cittadini, che non sono diverse a seconda dell'appartenenza politica; anzi forse mai come in questo momento, dal Nord al Sud, dagli imprenditori agli operai, tutti hanno un'unica esigenza: riportare il lavoro e la produzione al centro della discussione. E al riguardo penso al discorso di incentivare la spesa, una spesa che produce in Italia posti di lavoro che può produrre riqualificazione. Sicuramente, se non fossimo legati alle leggi europee, sarebbe bello stabilire che soltanto elettrodomestici italiani, soltanto mobili italiani, soltanto imprese italiane siano coinvolti in questo processo; questo non lo possiamo fare, però possiamo dire ai nostri cittadini che ogni volta che compriamo un prodotto *made in Italy* diamo un posto di lavoro e ogni volta che compriamo un prodotto che ha l'etichetta del nostro Paese abbiamo sicuramente un cassintegrato in meno.

onorevoli cittadini, colleghi senatori, il provvedimento al nostro esame mira a favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, in conformità al diritto dell'Unione europea, intervenendo sia attraverso modifiche ed integrazioni all'attuale impianto normativo, sia mediante la proroga e il potenziamento dei vigenti meccanismi agevolativi. ci saremmo aspettati che sui punti più qualificanti del provvedimento (in particolar modo mi riferisco agli articoli 14 e 16) vi fosse stata una maggiore possibilità di confronto sulle proposte presentate sia in Commissione sia in Aula; ce lo saremmo aspettati innanzitutto perché tutti sappiamo che ridurre le emissioni di gas serra, innalzare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e diminuire i consumi energetici in estrema sintesi è il contenuto del cosiddetto Pacchetto clima-energia 20-20-20 varato dall'Unione europea con l'obiettivo di contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili tramite obiettivi vincolanti per i Paesi membri. Poco prima del Protocollo di Kyoto, i temi ambientali erano considerati una scelta alternativa, assolutamente secondaria rispetto all'indirizzo comune. Oggi invece l'orientamento espresso dalla comunità europea vede nello sviluppo delle tecnologie verdi, in particolar modo nell'edilizia, lo strumento principe per poter per poter raggiungere l'ambizioso obiettivo proposto dal Pacchetto clima-energia. Il nostro attuale patrimonio edilizio, edificato in gran parte negli ultimi cinquant'anni, non ha tenuto conto alcuno della necessità di contenimento dei consumi energetici. Ne deriva che il recupero di tali edifici appare indispensabile innanzitutto per l'ambiente, ma anche per i grandi costi, sempre più insostenibili, che famiglie e imprese stanno sopportando. Costruire in modo intelligente, sostenibile e innovativo significa quindi realizzare case autosufficienti dal punto di vista energetico. La strada da percorrere, è quella di indirizzare dapprima i progettisti e poi anche la committenza

da fonti energetiche tradizionali. La bioedilizia e le «case passive» in particolare rappresentano una vera e propria sfida per il futuro della società contemporanea, in un tempo in cui le risorse energetiche scarseggiano e le sostanze inquinanti, dovute alle emissioni climalteranti, aumentano. La parola «*vintage*» la dice tutta sulla tendenza al riutilizzo. Bisogna guardare, per questo, all'utilizzo di nuovi materiali da costruzione e nel caso in cui questi non si vogliano o non si possano utilizzare, il recupero dei materiali oltre ad un vantaggio non indifferente dal punto di vista economico, offra risultati originalissimi e personalizzabili: è ecosostenibile, non necessita di tempo, energia e costi rispetto a quello creato si può definire «il bello a poco prezzo». Riciclare non è sinonimo di povero, tutt'altro. Oggi come oggi, la comodità viene percepita solo se vi è il consumo indiscriminato della fonte energetica. Non deve essere così, perché lo spreco di risorse dovuto ad abitudini errate costa in termini sia monetari che di salute personale e del pianeta. Da una lettura dell'ultimo rapporto dell'Osservatorio nazionale dei regolamenti edilizi si evince che 1.003 amministrazioni comunali in Italia hanno modificato il proprio regolamento edilizio per introdurre gli obiettivi di efficienza energetica e ambientale per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Ritengo che ormai il percorso intrapreso si indirizzi sempre più verso il tema delle città intelligenti, le *smart city*, quindi il posto d'onore è dedicato al tema dell'edilizia sostenibile e, indipendentemente dalla posizione geografica dei luoghi, questo nuovo approccio progettuale dovrà cambiare il modo di costruire nei settori sia pubblico che privato. Secondo il Movimento 5 Stelle nella fase dell'esame degli emendamenti, quest'Assemblea non può non tenere in giusta considerazione le proposte volte alla promozione della bioedilizia, che fornisce adeguate risposte a esigenze private e pubbliche di riduzione dei consumi energetici e di diminuzione delle emissioni di anidride carbonica. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ricordiamo che la direttiva n. 2010/31/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 9 luglio 2012. A norma di questa direttiva gli Stati membri devono stabilire e applicare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi e per quelli esistenti, assicurare la certificazione della prestazione energetica degli edifici e prescrivere l'ispezione regolare dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento. La direttiva fa obbligo inoltre agli Stati membri di assicurare che, entro il 2021, tutti i nuovi edifici rientrino nella categoria dei cosiddetti edifici a energia quasi zero. Il provvedimento in argomento si prefigge, finalmente, di recepire la suddetta direttiva. Parliamo di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano un frangente tanto delicato per il nostro Paese. Si tratta di misure di grande rilievo, capaci di agire su significativi risparmi, intervenendo su un settore che ultimamente ha conosciuto forti crisi, prevedendo un regime di significative detrazioni fiscali. vi è il *bonus* mobili, inserito tra le spese detraibili per l'acquisto dei mobili per l'arredo dell'immobile ristrutturato, fino ad una spesa massima complessiva di 10.000 euro. Può, quindi, fruire della detrazione del 50 per cento per i mobili, fino al 31 dicembre 2013, chi ha avviato una ristrutturazione a partire dal 26 giugno 2012, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto-legge

Il settore interessato genererà un'azione migliorativa di interi agglomerati urbani nel rispetto del territorio, mettendo in condizioni le imprese edili di programmare con lungimiranza il rilancio. L'immobile oggetto della ristrutturazione, anche grazie all'alacre lavoro delle Commissioni riunite finanze e industria, avrà indubbi vantaggi, con grande sollievo delle aziende operanti nel comparto legno e arredo. Contemperiamo il rilancio con i vincoli di bilancio e le ristrettezze note. Occupazione e sviluppo economico sono vitali per il nostro Paese e si tramutano nella politica di coesione territoriale, che trae fondamento e legittimazione dalla Costituzione italiana

di una società di garantire il benessere di tutti i suoi membri, ridurre al massimo le disuguaglianze ed evitare la polarizzazione». Il tema dell'efficienza energetica deve rivestire un ruolo primario nel rilancio dell'economia e dell'intero Paese. Bisogna osservare che il nostro sistema produttivo, colpito da una crisi mondiale senza precedenti, con il provvedimento in esame sottolinea la possibilità di promuovere il rilancio dell'economia energetica ed ambientale. Alla luce degli emendamenti presentati, anche l'indotto avrà indubbi vantaggi, con sollievo di famiglie e imprese. Dobbiamo adeguarci agli *standard* europei e tale adeguamento deve consentirci di dare ossigeno vitale alla piccola imprenditoria. Implementare nuove politiche di sviluppo urbano significa tutelarci anche da rischi ambientali e tale deve essere il significato dell'attestato energetico. Gli edifici nuovi dovranno rispettare i requisiti e, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, essere sottoposti a una valutazione sulla fattibilità relativa all'installazione di sistemi di fornitura di energia da fonti rinnovabili, pompe di calore, sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento urbano e sistemi di cogenerazione. Gli edifici esistenti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, dovranno beneficiare di un miglioramento della loro prestazione energetica, in modo da poter soddisfare i requisiti minimi. Possono essere esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi, tra gli altri, gli edifici ufficialmente protetti (ad esempio, gli edifici storici) e quelli adibiti a luoghi di culto; gli edifici residenziali utilizzati per un periodo limitato dell'anno; i fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadri; gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione e, in particolari casi, anche gli edifici industriali e artigianali. Si tratta di migliorare e promuovere l'attività tecnologica delle industrie, sostenendo nel contempo le famiglie che si accingono a ristrutturare un immobile, tenendo presenti i vari annessi, senza gravare sui conti pubblici. Oltre ad aiutare le famiglie, si concede un'opportunità all'industria degli elettrodomestici, che è sempre tesa a rinnovare prodotti con prestazioni energetiche all'avanguardia, riguardanti lo stesso risparmio energetico. Tutto ciò significa mantenere viva la ricerca e ravvivare una fonte di lavoro. In sintesi, ritengo che questo provvedimento sia di vitale importanza, sia per l'ambiente, sia per vari settori commerciali che caratterizzano l'economia del nostro Paese.

credo che sia emersa in modo evidente da tutti gli interventi che mi hanno preceduto la bontà del provvedimento, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale arrivo a dire, anche dal punto di vista psicologico. Contiene infatti quei caratteri della certezza, della concretezza, della sostenibilità e della immediata esecutività di cui il Paese ha bisogno. L'articolato, nel recepire gli indirizzi contenuti nella direttiva comunitaria n. 31 del 2010 sulle prestazioni energetiche degli edifici, che pone fine alla prolungata procedura di infrazione attivata nei confronti dell'Italia sulla direttiva n. 91 del 2002, interviene in modo diretto nella crisi della produzione e dei consumi

di domanda potenziale, di trascinamento dei consumi interni e di sviluppo di altri settori: sto parlando del settore dell'edilizia e di tutti i settori che attorno a questo ruotano negli ambiti della costruzione di materiali, di tecnologie e di competenze Ciò avviene nell'articolato attraverso il sostegno alla riqualificazione di un patrimonio immobiliare che ormai risulta inadeguato, obsoleto e troppo costoso rispetto alla disponibilità oggi di tecnologie di tecnologie che consentono risparmi certi e misurabili nei consumi energetici delle famiglie e delle imprese; la conferma e il potenziamento delle detrazioni fiscali agli interventi migliorativi dell'efficienza energetica e di ristrutturazione e la leva strutturale per lo sviluppo delle imprese, che nel risparmio nei consumi energetici trova elemento fondamentale per il superamento del *gap* negativo di competitività di cui soffrono le aziende italiane. Le misure già attivate negli anni precedenti, a partire dalla detrazione fiscale del 36 per cento sulle ristrutturazioni degli immobili, introdotta dal Governo Prodi, fino ad arrivare alle più recenti, connesse agli interventi per il miglioramento energetico degli edifici, hanno costantemente confermato la propria efficacia come volano di crescita economica e non solo. Nel periodo 2007-2011, le detrazioni sugli interventi migliorativi delle prestazioni energetiche degli edifici hanno attivato 17 miliardi di investimenti. Mi chiedo: quanti posti di lavoro corrispondono? Quanta ricchezza in rivalutazione del patrimonio hanno prodotto? Quanti consumi hanno generato nelle famiglie dei lavoratori e degli imprenditori? Quante imprese artigiane, che molti di noi definiscono l'ossatura del nostro sistema produttivo, hanno sostenuto? Quanto lavoro e quanto reddito in nero hanno fatto emergere?

con questi incentivi che oggi andiamo ad approvare, si raggiungerà la riqualificazione del 7 per cento del patrimonio immobiliare del Paese. Ciò significa che esiste uno spazio espansivo della domanda di investimento quindici volte più grande di quella che soddisferemo entro la fine del 2013. Bisogna però essere anche consapevoli

troppo ravvicinata, stabilita nel 31 dicembre di quest'anno, all'eccessiva durata dei tempi per il recupero dell'investimento effettuato attraverso la detraibilità estesa su dieci anni

avere il tempo nella fase emendativa di recuperare la terza criticità di questo provvedimento, che sta nell'esclusione dei soci delle cooperative di proprietà indivisa. Queste cooperative sono state istituite dal legislatore per favorire l'accesso alla casa delle categorie meno abbienti. Oggi un'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle entrate le esclude dai beneficiari di queste detrazioni. Credo che questa sia un'iniquità che va recuperata, e abbiamo la possibilità di farlo. È una nota interpretativa, e quindi siamo nelle condizioni quanto meno di porre rimedio alla più grossa iniquità contenuta nel provvedimento.

*relatore*. Signora Presidente, soltanto poche parole. Ho preso buona nota di quanto hanno indicato i colleghi in questa ampia discussione.

Sono state fatte alcune osservazioni non dico negative, ma non eccessivamente positive nei confronti dei relatori che, secondo alcuni, si sarebbero dimostrati eccessivamente asserviti al Governo. Abbiamo cercato di indicare in tutti modi le manifestazioni della Commissione e, quindi, riteniamo di aver svolto pienamente il nostro lavoro.

da parte di tutti i Gruppi, abbia valorizzato l'importanza di questo provvedimento per gli interventi che in esso sono compresi, volti a valorizzare il patrimonio immobiliare del nostro Paese e a dare un contributo importante all'efficientamento energetico dello stesso. Ovviamente siamo in una fase di passaggio anche nel regime degli incentivi e comprendiamo bene il senso il Governo ha voluto attribuire a questo provvedimento dalle scadenze prossime, dentro un regime di proroga e di aumento dell'incentivazione,

e a favorire investimenti in questo settore. Ribadiamo - come abbiamo detto nella relazione iniziale e come tutti i Gruppi hanno sottolineato - la necessità che nei prossimi mesi, in un lavoro comune tra Governo e Parlamento, si riesca a creare le condizioni strutturali, normative e finanziarie affinché le misure che qui sono state prorogate possano diventare stabili e rappresentare un riferimento certo per famiglie, imprese e consumatori. Se lo faremo, anche con modalità modalità diverse e una maggiore gradualità, penso che renderemo strutturale uno degli incentivi che maggiormente ha riscosso il successo dei consumatori e ha contribuito con misure anticicliche a sostenere un settore fondamentale dell'economia del nostro Paese.

Grazie, Tomaselli e Sciascia, per il grande lavoro di squadra che hanno dimostrato di sapere svolgere. Nessun asservimento al Governo: siamo entrambi dalla stessa parte, nel senso che lavoriamo nell'interesse del Paese e cerchiamo di applicare al meglio anche le direttive europee, che poi hanno ricadute nella vita dei nostri cittadini. Nel corso dell'esame in Commissione sono stati approvati diversi emendamenti, che certamente - per il lavoro che tutti i componenti hanno svolto - si possono ritenere integrativi e migliorativi. Alcune questioni ancora essere definite al meglio e quindi sono certa che l'Assemblea saprà trovare le migliori risposte Il decreto-legge contiene alcune norme ordinamentali di recepimento della direttiva

alcune modifiche riguardanti la definizione di «impianto termico», riducendo anche gli oneri di tipo amministrativo per gli impianti di piccola taglia: taglia: ciò testimonia che il dibattito è stato il più ampio possibile. Sono stati approvati anche altri emendamenti finalizzati a coniugare le opportunità offerte dall'efficienza energetica con lo sviluppo della nostra industria nazionale nostra industria nazionale di materiali, di costruzioni, di tecnologia ecocompatibile e con la promozione dell'occupazione. Voglio segnalare in particolar modo (dipendendo anche questo dal Ministero dell'economia) che è stato accolto un emendamento finalizzato all'estensione del Fondo di garanzia - che con il «decreto del fare» ha avuto un ampliamento di dotazione finanziaria finanziaria - anche ai costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica a seguito di interventi di efficientamento. È stata confermata

di concentrare al massimo gli strumenti e le risorse in funzione anticiclica.

non riusciremo ad inserire dotazioni finanziarie in questo provvedimento, ma sanciremo il principio, recependo un comma dell'emendamento che individua proprio la prevenzione, in materia di norme antisismiche, e demandando alla legge di stabilità Infine, voglio ricordare che la stessa strategia energetica nazionale, in merito alle detrazioni fiscali, prevede di estendere nel tempo questa misura, introducendo una serie di correzioni e di miglioramenti, per renderla più efficace ed efficiente in termini di rapporto costi‑benefici: a ciò ci siamo attenuti e a ciò ci continueremo ad attenere. Tra i possibili miglioramenti, i principali riguardano una differenziazione della percentuale di spesa detraibile, commisurata all'effettivo risparmio generato dall'intervento, l'introduzione di parametri di costo specifico massimo ammissibile per tipo d'intervento (per evitare fenomeni di traslazione di una parte dell'incentivo nei prezzi dei prodotti) e la specializzazione dello strumento per efficientare il patrimonio edilizio rivedendo il perimetro attuale degli interventi ammessi, in modo da evitare la sovrapposizione con altri incentivi.

il divieto - mi piace chiamarlo così - di cumulo di incentivi non è esaustiva, ma siamo certi che con la massima collaborazione tra Governo e Parlamento intero si possa addivenire a una realtà complessiva dove tutto il sistema viene aiutato e incentivato e non ci siano casi di sovrapposizione di incentivi su determinate tipologie energetiche, cosa che attualmente ancora permane.

alcune risposte che ancora lì non erano pervenute.

1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerando che le disposizioni ivi previste riguardano le materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea», "sistema valutario, sistema tributario e contabile dello Stato",

le materie "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e "tutela della salute", riconducibili alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: - all'articolo 5, comma 1, capoverso "articolo 4-*bis*" nel comma 2, appare opportuno che il decreto interministeriale ivi previsto, volto a definire il piano di azione destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia «quasi zero», sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, piuttosto che con il semplice parere della stessa; all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, capoverso "5-*quinquies*", si ritiene necessario che la norma ivi prevista sia formulata come facoltà, e non come obbligo, al fine di rispettare le competenze regionali in materia, con particolare riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale per lo svolgimento di attività di ispezione sugli impianti termici; - all'articolo 17, comma 1, capoverso 2, la norma ivi prevista appare invasiva della competenza costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali in materia di formazione professionale, in quanto configura un obbligo ad attivare un programma di formazione per tecnici installatori. Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: - sull'emendamento 8.6 parere contrario, in quanto il richiamo a materie riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato rende superflua la previsione di un obbligo di adeguamento regolamentare da parte di Regioni ed enti locali, dal momento che, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva spetta allo Stato, salva delega alle Regioni; sull'emendamento 12.4 parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, riguardando materia di competenza concorrente, sia formulata come facoltà e non come obbligo, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia; sull'emendamento 16.45 parere contrario, dal momento che la disposizione, nel limitare la detrazione di imposta ivi prevista alle sole coppie legate da un rapporto di coniugio, peraltro esclusivamente in base a matrimoni contratti dal 1° gennaio 2013, appare irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza; - sull'emendamento 16.0.7 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste appaiono lesive delle competenze delle Regioni e degli enti locali, oltretutto imponendo obblighi di natura onerosa, in violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta a Regioni ed enti locali dall'articolo 119 della Costituzione; sull'emendamento 17.201 parere contrario, in quanto finalizzato a trasformare da facoltà in obbligo il riconoscimento, a carico delle Regioni, di crediti formativi e ad introdurre ulteriori obblighi in tema di percorsi formativi,

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che: - dall'articolo 3 non derivino oneri aggiuntivi in capo alle amministrazioni pubbliche; in riferimento all'articolo 5, capoverso "Art. 4-*ter*", comma 2, lo stanziamento sul Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione dì reti di teleriscaldamento sia effettivamente adeguato a finanziare anche i progetti, di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, considerato peraltro che, secondo l'amministrazione competente, tale Fondo non è stato ancora attivato e non sono disponibili i dati statistici relativi alle escussioni effettuate; con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: - all'articolo 18, comma 1, deve essere espunto dall'elenco delle abrogazioni il riferimento all'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2005, posto che esso viene interamente sostituito dall'articolo 10 del provvedimento in esame e che, nella nuova versione, reca la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa; con la seguente osservazione: - si rileva che, secondo le amministrazioni competenti, le attività previste dagli articoli 8, 12 e 17, comma 2, possono essere effettivamente svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta sospeso l'esame degli articoli 14, 16 e 21». l'esame degli articoli 14, 16 e 21». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, in relazione alle parti precedentemente sospese, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: le coperture recate dall'articolo 21, comma 3, lettere *b)* ed *e)*, risultando a valere su risorse di conto capitale, potrebbero comportare una dequalificazione della spesa. Conseguentemente, non vi sono osservazioni sugli articoli 14 e 16». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.201, 5.11, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.204, 5.205, 6.14, 9.1, 9.4, 9.200, 13.0.1, 13.0.5, 13.0.5, 13.0.6, 14.1, 14.3, 14.5, 14.8, 14.10, 14.14, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.24, 14.25, 14.27, 14.30, 14.32, 14.36, 14.37, 14.38, 14.40, 14.41, 14.200, 14.201, 14.202, 14.203, 14.204, 14.300, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 15.3, 15.5, 15.9, 15.11, 15.200, 15.201, 15.0.1, 15.0.200, 16.1, 16.4, 16.5, 16.3, 16.6, 16.11, 16.12, 16.13, 16.18, 16.19, 16.20, 16.30, 16.32, 16.39, 16.35, 16.38, 16.37, 16.41,

16.0.4, 16.0.6, 16.0.200, 17.0.1, 17.0.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.200, 20.3, 20.5, 20.7. 20.200, 20.0.4, 20.0.200, 20.0.201, 20.0.202, 20.0.203 e 21.1. Sull'emendamento 5.9, il parere è di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 5, capoverso "Articolo 4-*ter*", comma 2, dopo le parole: "è utilizzato", delle seguenti: "entro i limiti delle risorse del fondo stesso"; sull'emendamento 6.15, il parere è altresì di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "è utilizzato", delle seguenti: "entro i limiti delle risorse del fondo stesso". A rettifica dell'avviso precedentemente espresso, in relazione ai chiarimenti fomiti dal Governo, il parere sull'emendamento 16.24 (testo 3), è di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole da: "da considerarsi inclusi" fino al termine del periodo. Sulla proposta 16.28 il parere è altresì condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole da: "Conseguentemente" fino al termine dell'emendamento. Sulle proposte 14.29, 16.29, 6.207, 12.200, 12.201, 13.0.200, 13.0.201, 6.200 il parere è di semplice contrarietà. Sull'emendamento 7.10, il parere è di semplice contrarietà, con la seguente osservazione: nell'estendere una fattispecie di esenzione, la proposta emendativa deve essere adeguatamente coordinata con l'esistente normativa europea di riferimento, al fine di evitare riflessi negativi in termini di procedure di infrazione. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti».

Grazie, utile rilevarla perché riguarda un tema su cui vi sono grandi discussioni in questo momento. Mi riferisco al rapporto tra minori entrate volte all'incentivo degli investimenti e la modalità per coprire tali minori entrate e poi

a valere su risorse di conto capitale e potrebbero comportare una dequalificazione della spesa, è in espressa e diretta violazione della norma di cui all'articolo 17, lettere *a)* e *c)*, della legge n. 196 del 2009, che è di diretta attuazione dell'articolo 81 della Costituzione; quindi, è una norma quasi interposta perché copre ben 540 milioni di euro di minori entrate correnti con stanziamenti di parte capitale, con la motivazione data dalla Ragioneria generale

...con la motivazione che queste minori entrate mettono in moto investimenti privati e, dunque, ben si possono sostituire investimenti privati agli investimenti pubblici previsti dal bilancio dello Stato. Siccome, come lei sa, date le politiche di risanamento, le spese per investimenti pubblici sono state gradualmente ridotte, questo non può essere un ragionamento accettabile per una forma di copertura, né può essere sostituito ad un altro ragionamento che invece noi dobbiamo fare, e cioè che gli incentivi agli investimenti privati generano nuove entrate correnti (come quelle relative all'IVA) che devono essere valutate e contabilizzate in bilancio per coprire queste misure. Lo dico, signora Presidente, a futura memoria, perché, siccome tale questione sarà il centro della discussione politica di finanza pubblica nei prossimi mesi, credo che questa linea e questo indirizzo, oltre alla violazione esplicita dell'articolo 81 della Costituzione che stiamo compiendo, non possa essere assecondato.

Ne prendo atto. Nell'espressione del proprio parere la 5a Commissione permanente opera una valutazione tecnico-contabile sulle coperture dei provvedimenti e degli emendamenti. la Presidenza non può che prendere atto, come prende atto, ovviamente, di quanto affermato dalla senatrice Lanzillotta. Onorevoli colleghe e colleghi, la Presidenza, dopo aver attentamente valutato gli emendamenti presentati, ha riscontrato alcune proposte estranee all'oggetto della discussione. In particolare, l'emendamento 14.0.5 modifica il limite relativo al divieto di ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare nelle aree sismiche; gli emendamenti 16.18, 16.19 e 16.200 sono diretti ad introdurre ulteriori detrazioni per i soli territori colpiti da alcuni specifici eventi calamitosi, mentre le proposte modificative 16.42 e 16.43 estendono la detrazione per ristrutturazione anche all'acquisto di mobili ignifughi; l'emendamento 17.0.1, invece, di natura ordinamentale, reca l'istituzione del piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali. Risultano altresì estranei gli emendamenti 20.0.5, diretto ad innalzare il limite relativo al divieto di trasferimento e uso di denaro contante e di titoli al portatore, e 20.0.200, in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno di manifestazioni culturali, nonché le proposte 20.0.2, 20.0.4, 20.0.201 e 20.0.203, recanti modifiche di natura ordinamentale al regime tributario in materia di IVA ed al relativo sistema sanzionatorio. La Presidenza dichiara pertanto improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 14.0.5, 16.18, 16.19, 16.200, 16.42, 16.43, 17.0.1, 20.0.5, 20.0.200, 20.0.2, 20.0.4, 20.0.201 e 20.0.203.

il miglioramento dell'efficienza energetica ad un'indagine *a posteriori* sotto il profilo dei costi, nel senso che qualunque intervento di efficientamento energetico proietta la sua efficacia molto avanti nel futuro, potremmo dire indefinitamente, cioè fino a che non termina la funzionalità della struttura stessa.

quando si ha un cambiamento di titolarità, perché quando cambia la titolarità, o per possesso o per fruizione, il locatario o l'acquirente prende in carico anche l'onerosità

di pensare di andare a cercare energia fuori, diversificando, bisognerebbe dare priorità alla generazione di energia *in loco* da parte di un'abitazione, e non solamente contenere il suo consumo energetico.

di promuovere la cultura della responsabilità in tema di valorizzazione dell'acqua di rete, quindi di risparmio della risorsa idrica, anche ai fini di contenere i consumi energetici e lo smaltimento di materie plastiche e di vetro. non solo avrebbe un carattere educativo importante ma sarebbe un segnale molto forte.

Quindi, si tratta solo di fare chiarezza normativa al fine di non compromettere la fattività delle norme delineate nel provvedimento. In particolare si prevede in primo luogo, in riferimento alla definizione di «cogenerazione» e di «cogenerazione ad alto rendimento», il richiamo esplicito alla normativa istituita, facendo capo al decreto legislativo 8 febbraio 2007, La definizione così prevista, oltre ad essere più corretta dal punto di vista giuridico poiché si riferisce ad una direttiva comunitaria di cui il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. atto di recepimento, consente l'installazione della cogenerazione in quanto tale, così come previsto dalla direttiva comunitaria in corso di recepimento. In linea con questo approccio, finalizzato ad evitare il sovrapporsi di definizioni suscettibili di determinare interpretazioni lacunose e ambigue, l'emendamento propone di inserire anche per la definizione di energia da fonti rinnovabili integrata da quella di biomassa il riferimento alla definizione più aggiornata, ai sensi del decreto legislativo che apporta sostanziali arricchimenti della vecchia definizione prevista dal decreto legislativo. n. 387/2003, quali il riferimento alla frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, nonché il riferimento alla pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, impegna

Presidente, interverrò brevemente per dare il senso dell'emendamento 2.26, sul quale spero i relatori vogliano esprimere, insieme al Governo, parere favorevole. Viviamo, ahimè, in un Paese a sismicità elevata, come scopriamo quotidianamente: gli ultimi eventi sono quelli della Lunigiana; prima c'è stato il Pollino, poi l'Emilia-Romagna e l'Abruzzo, e potremmo andare indietro negli anni, fino all'Irpinia ed oltre.

con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici.

Grazie, Signora Presidente, stante la sostanziale riformulazione dell'emendamento 2.1, ne chiederei il momentaneo accantonamento perché lo si possa verificare e decidere, sulla base del testo,

utilizzate per brevi periodi, come sono quelle che si trovano in località di villeggiatura, siano tenuti a sopportare nuovi oneri e costi in un periodo di grave crisi del settore immobiliare come quello attuale.

il parere contrario

aperta la votazione.

poiché sono molti vantaggiosi; servirebbero tra l'altro a rimuovere i problemi che si pongono all'esercizio delle reti elettriche e massimizzano il contributo che possono offrire alla compensazione mensile

Signora Presidente, al solo fine di agevolare i lavori, posso dirle che ad una

Dichiaro aperta la votazione.

M5S).* Le regole sono conosciute da tutti e valgono per tutti. Nessuno può votare per qualcun altro.

non ho fatto questo ritiro, e chiedo la votazione

Dichiaro aperta la votazione.

Signora Presidente, proprio in linea con quanto questo Gruppo ha sempre sostenuto nell'ultimo periodo riguardo alla questione dell'esclusione

e Province con finalità di miglioramento dell'efficienza energetica nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2013-2015. questione mira a favorire la realizzazione di nuovi edifici ad altissima prestazione energetica, in linea con quanto stabilito dalla direttiva europea 2010/31/UE.

Scopo dell'ordine del giorno è darci dei tempi. Vogliamo finalmente definire in quanto tempo programmiamo di ristrutturare tutto il patrimonio edilizio italiano, pubblico e privato.

Quindi, se il comparto edile è bloccato, sarebbe bene pensare di sbloccarlo invece di fare nuove costruzioni, cosa che il Movimento 5 Stelle ritiene inutile, cercando di ristrutturare l'esistente. Quindi, il senso dell'ordine del giorno è proprio questo: rimettiamo in moto il comparto edile, che ne ha bisogno, ma ristrutturando il tutto. Diamoci dei tempi: lo scopo è prevedere una politica che, entro vent'anni, ristrutturi tutto il parco immobiliare pubblico e entro venticinque ristrutturi tutto il parco privato. Rimettiamo in moto l'Italia, se ne siamo capaci.

Con tale emendamento chiediamo che vengano escluse dal Patto di stabilità le spese sostenute dai Comuni per gli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, che consente anche il potenziamento della sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento luminoso, nonché la messa a norma degli impianti.

Lanzillotta, la quale ha affermato che il Movimento 5 Stelle ha votato contro alcuni emendamenti importanti nel caso delle mozioni sulle partecipazioni statali. Questo non è vero, Resoconto stenografico alla mano, quindi chiediamo alla Presidenza di far rettificare alla senatrice Lanzillotta quanto esposto durante quella trasmissione.

stanchi, ma vorrei che chi ha chiesto la parola possa intervenire con calma. AIROLA *(M5S)*. Grazie, Presidente. Venerdì si è udito l'ennesimo grido di morte del mondo della cultura e dei beni culturali. hanno creato forte disagio al turismo: da Pompei alla Galleria degli Uffizi a Firenze. Tra sindacati (CGIL, CISL e UIL), l'UNESCO e il Ministero dei beni culturali sono intercorse critiche reciproche e accuse. Chi paga è in realtà l'intero Paese, perché il vero problema non è solo nella centrale e locale malagestione del patrimonio, non è solo nello sfruttamento dei lavoratori per gli organici sempre più esigui o per quelle cooperative appaltanti

è nell'assenza di una volontà di investire con un piano strategico sulla cultura. La colpa di questo e dei Governi precedenti è di aver ignorato la possibilità di concentrare investimenti e risorse nel più grande patrimonio artistico del mondo, nell'averci privato di un'economia florida e di un benessere economico e sociale e della possibilità di crescere in armonia e di evolverci in una società più giusta. La cultura è tutto questo. Ora, come abbiamo già fatto durante la discussione del DEF, ribadiamo che è imperativo stabilire un piano di investimenti ragionato e di rilancio di tutto il comparto cultura. Abbiamo già ricordato a quest'Aula e a voi senatori il numero impressionante di posti di lavoro e il rilancio economico di cui godrebbe tutto il Paese; e se aveste veramente a cuore questo Paese, dovreste attuare immediatamente queste istanze, altrimenti avremo l'ennesima conferma che preferite distruggere e svendere la nostra storia e permettere che l'ignoranza svilisca il popolo italiano rendendolo misero e succube. Gruppo M5S)*. Se siamo in quest'Aula oggi è anche grazie alla cultura che abbiamo ricevuto. Se voi senatori siete qui è grazie alla scuola e all'istruzione, i nostri beni. Vi prego di ascoltare il grido della cultura.

ha informato le organizzazioni sindacali, con una lettera raccomandata, dell'avvio formale delle procedure per 854 dipendenti in Italia. Solo in Piemonte (Regione da cui provengo e luogo di elezione) sono 267 i lavoratori che saranno messi in mobilità. Teniamo conto che parliamo in gran parte di donne di livello impiegatizio, nella totalità dei casi sprovviste di ammortizzatori sociali e che quindi, di fronte ad un mantenimento di questa procedura da parte della TNT,

non ci sono gli ammortizzatori. Questo è un altro durissimo colpo all'occupazione in questo Paese, e credo che convenga smettere, da parte del Governo,

veramente una preghiera in tal senso - che il Ministero dello sviluppo economico non gestisca in maniera burocratica questi fatti. La vicenda TNT è la punta di un *iceberg*, ma è un *iceberg* piuttosto grande.